il Presidente del Consiglio dei ministri ha inviato la seguente lettera: «Roma, 24 settembre 2021 Gentile Presidente, informo la Signoria Vostra che il Presidente della Repubblica, con proprio decreto in data odierna, adottato su mia proposta, sentito il Consiglio dei Ministri, ha nominato il prof. avv. Federico FRENI Sottosegretario di Stato per l’Economia e le finanze. F.to Mario Draghi». Comunico che in data 27 settembre 2021, è stato presentato il seguente disegno di legge: dal Presidente del Consiglio dei ministri e dai Ministri dell’economia e delle finanze, dello sviluppo economico e della transizione ecologica: Conversione in legge del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, recante misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale (2401) previ pareri delle Commissioni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

per cui si debba avallare l’idea che un’azienda statale possa applicare non il contratto collettivo nazionale, ma un regolamento interno al ribasso, peraltro

molto importante anche per il territorio romano, ma il tema è che questo è probabilmente un disastro economico, con un piano industriale inesistente e, in pratica, fatto al contrario, pieno di esuberi. MALAN

interstiziale acuta, specialmente tra gli anziani, cioè proprio nella popolazione più colpita da questa malattia. Va detto che l’Italia è il Paese con il più alto tasso di letalità (cioè del rapporto tra decessi

potrebbero anche essere legate insieme, quindi chiedo al Ministro cosa urgentemente intenda fare, perché in questo Paese c’è il rischio che le terapie che vengono date, a scapito di altre che sono state ostacolate in tutti i modi, causino un aumento dei morti, al contrario di quello che dovrebbero fare. Con l’occasione, sollecito anche una risposta all’interrogazione 405583, a proposito della questione della miopericardite. L’Italia ha dati straordinari: secondo le pubblicazioni dell’Aifa, ci sono soltanto due casi per milione di vaccinazioni che portano miocardite o pericardite. Guarda caso, in Israele i dati sono di 55 casi e negli Stati Uniti tra i 20 e i 50; in Italia, a quanto pare, abbiamo una popolazione fortissima, che non ha questo problema. Forse c’è un problema di rilevamento di queste reazioni avverse. Sollecito anche una risposta più che doverosa, come le altre peraltro, all’interrogazione 4-05137 del 24 marzo, in cui denunciavo il fatto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ora divenuto delle infrastrutture e